però, in Commissione bilancio vi è stata la certificazione di come quel patto c'è sempre stato, ma che è fragile e debole. Oggi il patto

dalla fiscalità generale alla copertura di un taglio del canone RAI, dà il senso dell'improvvisazione con cui questo Governo va avanti, ma anche della convinzione, per il Governo, che 400 milioni siano più utili per coprire un patto di potere, anziché per finanziare le liste d'attesa, che vanno ridotte e che continuano ad essere un problema per il Paese. *(Applausi)*. Questa vicenda si è risolta con un voto che ha visto il Governo essere battuto,

In questo decreto-legge chiediamo che si intervenga su un altro strumento di finanziamento del sistema sanitario, perché il Governo non lo finanzia in maniera adeguata; facciamo facciamo riferimento alla necessità, già evidenziata in Conferenza delle Regioni praticamente da quasi tutte le Regioni, di intervenire sui meccanismi di controllo della spesa farmaceutica (ci riferiamo al *payback*) chiediamo davvero di aprire un dibattito serio, a margine del confronto sul fisco, su come le leve fiscali debbano finanziare alcuni servizi indispensabili, a partire dalla sanità pubblica. Signora Presidente, chiudo chiedendo, in alternativa, di anticipare anche i tempi della Conferenza dei Capigruppo e di fermarci qui, perché avremmo dovuto votare gli emendamenti di un altro provvedimento. Penso che abbia molto senso che i Presidenti dei Gruppi si confrontino urgentemente per decidere l'andamento dei lavori.

Signor Presidente, condivido l'analisi che il presidente Boccia ha appena fatto. Sono membro della Commissione bilancio, quindi ho potuto apprezzare tutti i lavori di queste giornate inutili: abbiamo iniziato a votare questa mattina il provvedimento ma gli emendamenti erano stati depositati due settimane fa e i pareri del Governo ancora oggi sono lacunosi, tanto che dopo settimane di discussione ci sono degli emendamenti ancora accantonati rispetto ai quali il Governo si rimette alla Commissione e il relatore non sa che parere esprimere perché non ha il parere del Governo. Siamo quindi in una situazione paradossale in Commissione bilancio: siamo bloccati dalla maggioranza per colpa della sua litigiosità, di cui mi interessa il giusto, perché è del tutto evidente che questa maggioranza, come sempre il centrodestra fa, sta insieme per poter esercitare dei piccoli spazi di potere, ma non ha una visione comune del Paese. Questo mi preoccupa perché, per colpa di questa litigiosità, vi sono degli elementi di risposta ai problemi dei cittadini, anche quelli molto più banali rispetto a quelli citati dal presidente Boccia, che potrebbero avere risposta anche in questo provvedimento, ma che, per la tensione che c'è tra i Gruppi di maggioranza, non si riescono a fare. Penso ad esempio alla risoluzione del problema delle quote latte: un emendamento di buon senso, riformulato da parte del senatore Bergesio, esce dal dibattito perché non c'è confronto tra i Gruppi di maggioranza.

in questa maggioranza, esso debba essere chiarito all'interno delle forze che la compongono, ma questo non può essere un elemento che va a detrimento della capacità del Parlamento di dare risposte ai cittadini. Questa è la parte più grave di quello che sta accadendo. Se c'è una crisi di maggioranza - lo ripeto - me ne importa il giusto; a me interessa che questa crisi non imponga un percorso falsato in Commissione, dove si possono fare delle cose per dare tutele a chi non ne ha. la mia richiesta è di anticipare il prima possibile la Conferenza dei Capigruppo e di non iniziare con le votazioni sul decreto-legge sul numero chiuso a medicina. Prima di ricominciare i lavori in Commissione bilancio e le votazioni in Aula, chiedo di riunire la Conferenza dei Capigruppo. Signor Presidente, un'Assemblea parlamentare funziona con i voti. Al di là delle considerazioni un po' speciose o strane che ho sentito in questi due interventi sull'ordine dei lavori, vorrei ricordare l'aspetto pratico di certe votazioni. Nella votazione che si è appena tenuta in Commissione bilancio in realtà l'aspetto pratico è molto semplice, vale a dire che chi in questo momento ha parlato di fiscalità generale e di cose di questo tipo ha semplicemente detto di no a uno sconto di 20 euro per 20 milioni di italiani e 20 milioni di famiglie. Tutto qui, si è deciso di far pagare di più, quindi di aumentare le tasse per 20 milioni di cittadini. Basta che si sappia, senza dover andare a trovare chissà che motivazioni, perché vede, senatore Boccia, non è che c'è una tasca che si prende questi soldi della fiscalità generale e se li intasca. Questi soldi della fiscalità generale - per il tramite del Presidente invito il senatore Boccia a prendere nota di ciò che evidentemente non ricorda dai suoi studi - sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei cittadini e invece vengono prelevati. Basta che si sappia. Chi fino a adesso ha parlato di sconti, di sgravi ai cittadini e di cose di questo tipo ha semplicemente votato per far pagare 20 euro in più a 20 milioni di cittadini. Tutto qui. Per il resto, chi ha deciso di sostenere questa scelta delle opposizioni evidentemente avrà avuto le sue motivazioni. Dovrà poi spiegarlo, come tutti, come anch'io spiego sempre ogni mio voto ai cittadini. Non c'è nessun problema e non capisco che tipo di dramma ci sia se ogni tanto in Parlamento - vivaddio - si mettono in chiaro le posizioni di chi vuole fare chi e che cosa, perché questo è ciò che secondo me dovremmo fare un po' più spesso, senza drammatizzare e altre scene di questo tipo. Ci sono dei voti e ogni voto ha un suo significato. La Lega è sempre stata contro il canone RAI, è sempre stata per avere meno tasse per i cittadini e sempre lo sarà. Noi continuiamo a difendere questa impostazione.

la vicenda che si è appena consumata all'interno della Commissione bilancio ha un inevitabile impatto di carattere politico e di natura procedurale sui nostri lavori. Siamo dell'opinione che non si possa mettere tra parentesi questa vicenda e che occorra immediatamente procedere alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo, senza indugio e senza aprire la discussione e le votazioni sul provvedimento all'ordine del giorno, perché la questione va ben oltre l'elemento in sé, che è già un elemento impegnativo dal punto di vista dell'impatto popolare e dell'equilibrio politico. Sull'equilibrio politico la lettura è molto semplice: la Presidente del Consiglio ha ritenuto di dover assecondare la posizione di un suo alleato, la Lega, contro la posizione di un altro suo alleato, Forza Italia. *(Applausi)*. che stanno iniziando una serie di segnali di fumo, di *ballon d'essai*, di messaggi incrociati all'interno della maggioranza, in vista probabilmente di una resa dei conti che non si circoscrive esclusivamente a quello che è accaduto questa mattina. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo chiudere gli occhi quantomeno su tre fenomeni macroscopici di rottura all'interno della maggioranza, che impongono una riflessione di carattere generale. Senza entrare nel merito di vicende che sono decisamente poco commendevoli e che abbiamo letto oggi sui giornali, quelle di uno scontro interno al partito della *Premier* sulle nomine, noi stiamo assistendo in queste ore ad uno scontro profondo tra la Lega e Forza Italia sul tema dell'assetto bancario, del futuro delle banche italiane e di operazioni di mercato che sono state annunciate. *(Applausi)*. E tremiamo all'idea - se posso permettermi che il vice premier Salvini si applichi sulle banche con la stessa dovizia con la quale si applica sui trasporti del nostro Paese. *(Applausi)*. Ma su questa vicenda, che è una vicenda delicatissima, la maggioranza è spaccata. La maggioranza è spaccata anche su un'altra questione, che si annuncia, che si riverbera, che preoccupa. Si annuncia l'emanazione da parte del Governo di un decreto-legge, l'ennesimo, che interviene in materia di giustizia e in materia penale sulla questione della *cybersecurity* e si dice

spaccatura all'interno della maggioranza; Forza Italia, da una parte, e il resto della maggioranza, dall'altra. Oggi, mentre noi siamo qui, si sta compiendo la spaccatura politica più clamorosa agli occhi di tutta Europa.

è solo un'anticipazione e una fuoriuscita di un tema strutturale molto più profondo, che impone dal punto di vista politico una riflessione e, dal punto di vista procedurale, un'immediata ricalendarizzazione dei nostri lavori.

di ostruzionismo di maggioranza, chiamiamolo così. Ha fatto bene - e mi associo a questa considerazione - il presidente Boccia a chiedere il ritiro del provvedimento. Capisco che da parte dei colleghi di maggioranza ci sia un tentativo di minimizzare quello che sta accadendo. di maggioranza ci sia un tentativo di minimizzare quello che sta accadendo. Mi pare però che questo tentativo di minimizzazione non faccia i conti con la realtà. Peraltro da molte settimane, da molti mesi a questa parte,

delle principali riforme che avete portato avanti, cioè la scellerata autonomia differenziata e, guarda caso, da quando è successo, si è inevitabilmente dovuta bloccare l'autonomia differenziata e sono arrivati *stop* su vari provvedimenti. Si sta sgretolando il patto attorno al quale avevate costruito la tenuta della maggioranza, quel famoso scambio politico che noi forze di opposizione denunciamo da molti mesi a questa parte. Penso che la paralisi che sta avvenendo in questi giorni e in queste ore nei rami del Parlamento, abbia anche molto a che fare con il fatto che fin quando non si capisce come procederanno i principali provvedimenti della maggioranza parlamentare - l'autonomia differenziata, da una parte, e il premierato, dall'altra e il premierato, dall'altra - ci sarà la guerriglia alla quale assistiamo tutti i giorni. Sono tutte cose comprensibili dal punto di vista politico, peccato però che questa guerriglia e questa paralisi incidano direttamente sul Paese. Anche in questo caso, non fate propaganda a basso costo. Parliamo seriamente anche della vicenda del canone della RAI. Davvero qualcuno può sostenere ragionevolmente che l'operazione di propaganda portata avanti in maniera così smaccata e così clamorosa

si recuperano naturalmente dalla fiscalità generale, in un Paese in cui, come sappiamo, le tasse le pagano soltanto in pochi *(Applausi)* e le pagano sempre e solo i lavoratori dipendenti, perché una parte consistente del Paese continua purtroppo ad evadere. Anche vogliamo fare davvero una riflessione sulla RAI, senza propaganda? Vogliamo farla davvero una riflessione sulla RAI intesa come servizio pubblico, come bene comune? Ma davvero pensate che un tema grande come quello della della RAI come servizio pubblico e come bene comune si possa affrontare semplicemente con un'operazione così smaccatamente propagandistica? Se ne vogliamo parlare seriamente, facciamolo, ma davvero evitiamo la propaganda a basso costo, quella degli 1,67 euro al mese, presentati per l'appunto come una grande riforma ma poi recuperati in un altro modo, dalla fiscalità generale. Dalle parti mie, questo si chiama gioco delle tre carte e fin quando lo si fa in qualche in qualche strada del nostro Paese, ancora ancora, fa anche sorridere, ma francamente quando lo si fa in Parlamento davvero sconcerta.

al provvedimento ancora non adottato sulla giustizia e sui poteri della magistratura e delle realtà investigative, al decreto sulla RAI, quindi potremmo parlare per ore sull'universo mondo e portare altri argomenti a piacere. Comprendo gli interventi dell'opposizione, probabilmente a ruoli invertiti avrei fatto gli stessi interventi, quindi non mi meraviglio assolutamente, ognuno deve fare la sua parte. che la maggioranza è assolutamente operativa e coesa su tutti i provvedimenti. Lo vedremo tra qualche minuto quando sarà varato un provvedimento ampiamente atteso dal Paese quale quello che riguarda l'accesso alla facoltà di medicina e ringrazio fin d'ora il ministro Bernini che vedo disciplinatamente al suo posto per questa misura che riguarda le famiglie,

dal senatore Boccia; l'esame del provvedimento è andato avanti e poco fa è stato prorogato il concordato fiscale, che porterà soldi allo Stato e vantaggi alle imprese e alle famiglie. Votatele queste misure, invece di fare lo *show* intorno ad altri argomenti. Quindi, noi andiamo serenamente avanti sui temi della giustizia, delle riforme, del fisco, dell'economia, della legge di bilancio e anche dell'Unione europea, dove l'Italia avrà un Vice Presidente esecutivo che i vostri Governi non hanno ottenuto

con l'impegno della Presidente del Consiglio, del vice presidente Tajani, del Partito popolare europeo, dei conservatori e di tutti quelli che hanno visto, con la designazione di un Vice Presidente esecutivo, un successo italiano che altri non hanno avuto. Se poi volete parlare dei poteri della super procura antimafia, ne parliamo quando volete, anche in Aula. Noi aspettiamo ancora che persone come Cafiero De Raho decidano se stare in Commissione antimafia, visto che li convoca la procura della Repubblica di Perugia. *(Applausi)*. È stato convocato dalla procura della Repubblica di Perugia, quindi fanno tutto loro. Per quanto riguarda il canone, se vi interessa, la posizione del Gruppo Forza Italia non è nuova. non è nuova. Comprendo la posizione dei colleghi, che rispetto e con i quali ho discusso, ma si sta discutendo se portare da 90 a 70 euro il canone della RAI, che si traduce in 50 centesimi a italiano al mese e in 1,6 euro a famiglia:

lo Stato, come è successo l'anno scorso, deve dare 430 milioni di soldi pubblici alla RAI. Noi riteniamo che sia una partita di giro. Da un lato il singolo cittadino ha un piccolo vantaggio, poi il

Tutto qui. Abbiamo un punto di vista che esprimiamo da tempo, sul quale abbiamo mantenuto una posizione; non siamo d'accordo, non è su questo che si fonda il patto di Governo. Il patto di Governo si fonda anche sul taglio delle tasse che noi faremo con il cuneo fiscale, che è finalizzato ad aumentare il reddito reale. Votate a favore di queste misure! Voi, invece, votate contro il reddito delle famiglie e fate gli scioperi con i vostri sindacati quando l'occupazione cresce e la disoccupazione cala. cala. La maggioranza c'è, voi avete sperperato soldi con il reddito di cittadinanza e con i *bonus* non finanziati; la maggioranza c'è e ha la propria libertà di

che noi abbiamo votato per la nostra posizione, è lui che ha votato con noi. Se loro votassero sempre come Forza Italia, si troverebbero meglio e sosterrebbero il Governo Meloni insieme a Forza Italia.

taglio del cuneo fiscale, più occupazione e altri interventi. Voi votate per le tasse, mentre noi le tasse le tagliamo. Buon lavoro.

una nuova finestra"). Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario vigente e il nuovo calendario dei lavori fino al 9 gennaio. Nella seduta di oggi proseguirà, fino alla sua conclusione, l'esame del disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di medicina e chirurgia. Domani, a partire dalle ore 9, avrà luogo la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un senatore Segretario. Dopo la chiama le urne rimarranno aperte fino alle ore 12. Alle ore 11 saranno esaminati rendiconto 2023 e bilancio interno 2024 del Senato. Seguirà la discussione del decreto-legge in materia di misure economiche e fiscali. Secondo quanto anticipato dal Governo, si è stabilito che, dopo la posizione della questione di fiducia, si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. Il sindacato ispettivo e il *question time* già previsti per domani non avranno luogo. Nella settimana dal 3 al 5 dicembre saranno discussi i decreti-legge su lavoratori stranieri e flussi migratori e in materia di tutela ambientale. anticipato dal Governo, si è stabilito che, dopo la posizione della questione di fiducia, si passerà per ciascuno dei provvedimenti direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. Giovedì 5 dicembre, alle ore 15, avrà luogo il *question time*. Nella settimana dal 10 al 12 dicembre saranno discussi i seguenti argomenti: legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023; disegno di legge su libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare; disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, in materia di lavoro; istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario. Giovedì 12 dicembre, alle ore 15, avrà luogo il *question time.*

Nella settimana del 16 dicembre, che prevede sedute senza orario di chiusura fino a sabato 21, se necessario, saranno discussi il decreto-legge in materia di lavoro, università e PNRR e il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2025. L'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati. A tale riguardo, sono previste sedute senza orario di chiusura anche nella settimana dal 23 al 28 dicembre. Mercoledì 18 dicembre, alle ore 10, si terrà la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2024. Il testo delle comunicazioni stesse, dopo l'illustrazione presso la Camera dei deputati, sarà consegnato in Senato dalla presidente Meloni martedì 17, orientativamente intorno alle ore 11. Dopo le festività di fine anno, l'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 8

internati italiani nei campi di concentramento e della cittadinanza digitale, nonché, ove concluso dalle Commissioni, con la discussione del disegno di legge in materia di morte medicalmente assistita. Giovedì 9 gennaio avranno luogo il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*. Il calendario potrà essere integrato con deliberazioni concernenti proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di attivazione di conflitti di attribuzione.

Signor Presidente, vorrei chiarire il perché del nostro voto contrario

di prevedere che ci sia una programmazione del fabbisogno di medici in base al fabbisogno di salute della popolazione. Per queste ragioni siamo contrari all'abrogazione di questa parte della delega.

e su moltissime altre facoltà biomediche, con il ridisegnamento degli ordini degli studi di moltissime facoltà. Noi vorremmo che ciò sia fatto bene

norma che sia efficace e non debba costringere le università e gli studenti a una grande sofferenza organizzativa.

ci sia un semestre comune a diversi corsi di studi; poi sarà il Ministero a decidere quali sono i corsi di studi che verranno inseriti nel semestre comune. C'è un punto però da considerare: mentre oggi a medicina entrano 20.000 studenti, con la modifica si dovranno seguire in questo primo semestre circa 90.000 studenti; questi sono quelli che ogni anno provano ad accedere alla È chiaro che al momento - per come è il nostro sistema universitario - non ci sono né i docenti, né le aule, né sono state stanziate le risorse per fare questo. Allora, noi vediamo all'orizzonte un grande rischio e, cioè un'apertura alle lauree telematiche, cioè ai corsi di studio telematici che potranno venire in soccorso se non si riesce a rafforzare tutta l'infrastruttura che dovrà prevedere

va bene inserire e mettere in rete diversi corsi di studio, però escludiamo tutte le lauree telematiche. In Commissione il parere del Governo è stato contrario, con una motivazione che non può giustificare la contrarietà. La motivazione è che oggi le lauree in medicina non sono accreditate per le lauree telematiche. Non ci sono università telematiche con l'accreditamento per medicina. Il punto, però, è che, facendo un semestre comune a diversi corsi di studio, rientreranno tutte quelle università telematiche che invece hanno l'accreditamento, per esempio, per biologia, per farmacia, per biotecnologia. Non sappiamo quali saranno i corsi affini, ma c'è il rischio che corsi telematici accreditati per altre discipline scientifiche possano entrare. Allora, aver bocciato questa proposta significa tradire - a nostro avviso - un'intenzione. Passo all'emendamento 2.101,

Come verrà fatta la nuova graduatoria per l'accesso a medicina? Verrà fatta in base al superamento degli esami del primo semestre. Per noi è fondamentale che non siano i singoli docenti a dare un voto per il superamento, ma siano dei test nazionali; altrimenti succederà che ci sarà troppa discrezionalità non solo tra università e università, ma anche tra docente e docente. Noi avevamo quindi chiesto di inserire che gli esami del primo semestre venissero fatti secondo *standard* nazionali e in forma scritta: per noi questo è un punto importante. Devo riconoscere che è stato inserito nel testo che si seguiranno degli *standard* nazionali, come noi chiedevamo; non è stato specificato che la modalità di svolgimento sarà in forma scritta. Per noi questo è importante, perché altrimenti davvero si rischia che sia il singolo docente a decidere chi debba avere un voto alto per entrare a medicina e chi no. Passo a un altro emendamento che affronta un altro punto critico del disegno di legge delega, che è quello delle risorse. L'emendamento 2.112 chiede che vengano stanziate risorse anche per garantire più più borse di studio e più alloggi universitari. Anche in questo caso riconosco l'impegno di ieri della Ministra che ha specificato in Aula che verranno stanziate risorse per riuscire riuscire a riconoscere il diritto allo studio a un numero maggiore di studenti. A nostro avviso, però, andava inserito già nella legge delega.

in parallelo. Tuttavia, a nostro avviso, andrebbe specificato un sostegno maggiore per gli ambiti di specializzazione carenti, ma spero che ciò verrà fatto con un successivo provvedimento.

prende in considerazione un problema che abbiamo sempre sottoposto al Governo, fin da quando ci siamo messi a lavorare su questi provvedimenti. Il punto è che possiamo anche occuparci della riforma dell'accesso a medicina, ma questa dovrebbe andare di pari passo con la riforma delle scuole di specializzazione,

anche in relazione alle singole aree di specializzazione. La Ministra sa bene - lo dico a chi ci ascolta - che in questo momento abbiamo in Italia un problema enorme, perché molti posti di alcune tipologie

a prevalente carattere teorico - chiaramente non possiamo far accedere 90.000 persone nei laboratori o a insegnamenti diversi da quelli teorici

in questo momento è che senza risorse, adeguati spazi e l'assunzione di nuovo personale, è impossibile accogliere 90.000 studenti nelle nostre università. La distribuzione fra vari corsi di studio è una soluzione adeguata. Può darsi che il Governo abbia in mente questa prospettiva e, quindi, ci chiediamo perché non avete voluto accogliere questo emendamento,

venisse approvato, sarebbe una garanzia per tutti quegli studenti che nel 2021 sono stati costretti dal Covid a stare in casa, davanti a un *monitor*, anziché andare a scuola. Come ho detto ieri, pensare anche lontanamente che una possibile soluzione per quegli studenti sia di seguire il primo semestre davanti a un *monitor* a casa sarebbe un disastro. Questo emendamento esclude questa possibile eventualità. Se è davvero nella volontà del Governo evitare che gli studenti non stiano davanti

che poteva essere riformulato sul semestre, anziché sul primo anno, come avevamo proposto noi. L'altro emendamento che vorrei sottolineare è il 2.123,

tutti i colleghi della maggioranza hanno detto che a un disegno di legge delega non vanno assegnate le risorse. Io sono alla prima legislatura e mi sono fidata.

nel prosieguo del ragionamento sulla organizzazione, saranno messe le adeguate risorse. Signor Ministro, se lei assicura questo, perché la sua maggioranza non approva questo emendamento che impegna il Governo a mettere le adeguate risorse? Forse solo perché l'ha proposto la minoranza? Ma io lo regalo alla maggioranza! Lo firmino loro questo emendamento e lo approvino!

Presidente, intervengo per spiegare perché votiamo contro questo emendamento. Noi pensiamo che dare più tempo per la legge delega sia un danno per gli studenti, che resterebbero, in questo caso, per due anni in attesa della riforma. Noi, invece, riteniamo che un anno debba essere più che sufficiente per dare certezza di quale sia il nuovo percorso di accesso.

qui c'è esattamente l'abolizione del numero chiuso, attraverso la soppressione di una serie di lettere dell'articolo. E c'è esattamente quella che è la battaglia storica dei movimenti studenteschi, dei collettivi, delle associazioni, cioè di tutti quelli che all'interno delle università in tutti questi anni - perché la battaglia contro il numero chiuso a medicina attraversa gli atenei italiani da molti anni a questa parte - ritengono - e secondo noi lo ritengono giustamente - che il numero chiuso è un drammatico strumento selettivo, peraltro profondamente classista, e chiedono di poter immaginare l'ingresso alla facoltà di medicina in un'altra maniera rispetto a come è accaduto in tutti questi decenni. Nell'emendamento naturalmente vengono previste delle coperture e soprattutto viene previsto un investimento strutturale, perché - e questo è il vero punto debole del vostro provvedimento, che non abolisce evidentemente il numero chiuso - questo non si può fare se non si incrementano i finanziamenti. Abolire il numero chiuso pensando che i finanziamenti restino gli stessi è impossibile. E infatti, questo vostro provvedimento, che - come sappiamo - è ad invarianza di bilancio, il numero chiuso non lo abolisce. Noi invece lo vogliamo fare: è una battaglia storica della mia forza politica e una battaglia che Alleanza Verdi e Sinistra sposa in pieno, quella per l'appunto dei gruppi studenteschi, dei movimenti e delle associazioni che da anni hanno dato vita a comitati che in tutta Italia lottano su questo. È un emendamento che perlomeno penso che consentirà di fare chiarezza. Non pretendo che tutti lo votino, perché so bene che sul numero chiuso ci sono pareri discordanti, ma pretendo e chiedo che ogni forza politica si prenda la responsabilità delle proprie azioni. Si può certamente essere a favore del numero chiuso - ed io non sono a favore del numero chiuso - ma l'unica cosa che non si può fare è dire che si è contro il numero chiuso e poi invece nella pratica continuare ad essere d'accordo. Anche questa riforma viene raccontata dalla stampa come l'abolizione del numero chiuso. Leggo gli articoli dei giornali: «Orizzontescuola» titola a nove colonne: medicina: addio a numero chiuso; un altro giornale: medicina, stop al numero chiuso. Ecco, non stiamo parlando di questo: stiamo parlando di altro.

lo abolisce. Chi non lo vota perlomeno ci risparmi la retorica.

la richiesta di reperire più risorse, dall'altro dire però che si abolisce *tout court* il numero chiuso e confondere il numero chiuso con il numero programmato è un grave errore. Abbiamo una direttiva europea che chiede a tutti gli Stati europei di programmare il numero di professionisti e di medici che operano in sanità in accordo al fabbisogno di salute della popolazione. Quindi l'Italia, come tutti gli altri Paesi europei, deve garantire una programmazione dei medici che ci saranno in futuro. Quello che abolisce questo provvedimento non è il numero chiuso, bensì l'attuale *test* di ammissione a medicina, mentre garantisce e continua a garantire una programmazione. A nostro avviso, chi conosce il sistema di formazione medica in Italia riconosce che c'è una qualità altissima, che noi non siamo disposti a barattare dicendo che si può accedere alle facoltà di medicina senza alcuna programmazione

la facoltà di medicina non deve essere appannaggio delle università telematiche e che il corso di studi in medicina e chirurgia non deve essere appannaggio delle università telematiche, questo emendamento noi chiediamo di specificare nel provvedimento che anche nel semestre comune, in cui verranno inseriti altri corsi di studio, che non sono solo quello di medicina, ma sarà biotecnologia, sarà farmacia - deciderà poi il Ministero quali sono gli altri corsi di studio - non si inseriscano le università telematiche.

parliamo di crediti formativi, cioè di esami - stiamo anzitutto ledendo la libertà di insegnamento e poi stiamo riducendo la didattica a una forma di test.

universitari, se lasciamo al singolo docente la discrezionalità di dare un voto per questi esami, da cui poi dipenderà l'ingresso alla facoltà di medicina, non solo rischiamo di creare una disparità da università a università e da docente a docente, ma poi - a nostro avviso - andiamo a rendere davvero complicata la creazione di una graduatoria nazionale. A nostro avviso invece, così come oggi oggi c'è un test nazionale, allo stesso modo ci dovranno essere più test nazionali per le varie discipline inserite nel semestre comune.

di avere accesso a università come Cambridge, Oxford e Imperial College, con un effetto democratizzante sull'istruzione.

del primo semestre. Noi riteniamo, invece, che in questa riforma importante che si sta facendo dell'accesso alle facoltà di medicina vadano inseriti anche i medici di medicina generale e tutti quei professionisti che operano sul territorio, anche perché, ampliando la platea a 90.000 studenti, è chiaro che non potranno fare da *tutor* solo i professori universitari, quindi bisogna utilizzare tutto il personale sanitario e medico a disposizione, anche quello sul territorio. la ragione di questo emendamento è il fatto che, di fronte a una pressione come quella che si realizzerà con l'aumento degli studenti, avremo bisogno di persone che conoscono la materia.

e noi lo stiamo chiedendo a dei medici di medicina generale, a dei medici ospedalieri che l'ultima volta che hanno aperto un libro di biochimica o di fisica risale praticamente a quarant'anni fa: qui stiamo raschiando il fondo del barile. Questo emendamento dimostra esattamente la situazione in cui ci troveremo. Vi state attaccando all'ultimo chiodo per poter fare questa cosa. Permettere ai medici di medicina generale, ai clinici degli ospedali di insegnare medicina ai nostri ragazzi del primo anno è irresponsabile.

questa lettera *n)* stabilisce una cosa molto strana per chi si occupa di scuola, perché parla di promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado,

relatore Zaffini. Il PNRR, nelle tante riforme che sono state fatte, ha portato un'importante riforma dell'orientamento, che il vostro ministro Valditara vanta e sbandiera ad ogni angolo; si dice che grazie a questa riforma del PNRR ci sarà la possibilità di orientare tutti i ragazzi, a partire dal triennio della scuola secondaria di secondo grado. dite che l'orientamento deve essere specifico per queste discipline e per questi indirizzi, dimenticandovi tutto il resto dell'orientamento, perché se aveste voluto potenziare necessariamente questo orientamento, avreste dovuto stanziare delle risorse. Se non ci mettete dei soldi, quelle risorse già a disposizione

se non altro a mettere un paletto dicendo: facciamo in modo che l'orientamento più specifico per questi indirizzi avvenga nell'ultimo anno e facciamo vedere a questi ragazzi come si lavora veramente lì dentro e prevedendo la possibilità di un tirocinio. Voi, invece, avete provato ad affrontare questo tema in maniera disordinata, perché quello che vi interessa è solo la bandierina ideologica da andare a rivendervi. Tuttavia, come vi è stato spiegato bene caso non solo non intervenite su un vero numero, su quello che serve ai percorsi di medicina, ve lo venderete come abolizione del numero chiuso (che non c'è) e, dall'altra parte, peggiorate anche la possibilità di un sistema di numero programmato. Voglio infatti vedervi, dopo i primi sei mesi, come regolamenterete la possibilità di accesso dei ragazzi che magari sono a pari con tutti i percorsi che voi state loro chiedendo. Ci sarà un bel caos, di cui voi sarete responsabili.

un altro era aver frequentato dei licei a curvatura biomedica. Nella versione originale di questo disegno di legge c'era quasi un ingresso diretto o comunque un ingresso riservato a tutti quegli studenti che avevano frequentato i licei a curvatura biomedica. biomedica. Questo chiaramente l'abbiamo modificato - e ancora una volta ringrazio il relatore in Commissione - perché avrebbe significato ridurre la platea e privilegiare tutti quegli studenti che vivono, per esempio, nelle grandi città in cui sono più diffusi i licei a curvatura biomedica, mentre chi vive in periferia sarebbe stato

non siano di quota superiore a un sesto rispetto al totale dei crediti, proprio perché riteniamo che, se si sbilancia troppo il credito a favore del liceo a curvatura biomedica, allora si rischia di escludere una platea importante

insiste su un tema fondamentale su cui molto ieri abbiamo discusso durante il dibattito generale. È stato anche uno dei temi centrali - lo sa la Sottosegretaria che ha seguito i nostri lavori nostri lavori - della nostra discussione in Commissione. Noi pensiamo che questa sia una falsa riforma: sia in realtà un tentativo di aggirare un'istanza giusta

Abbiamo denunciato la mancanza di risorse, come veniva detto: superare realmente il numero chiuso è possibile solo con investimenti a sostegno dell'offerta del Sistema sanitario nazionale; è possibile solo mettendo in condizione tutti gli studenti e le studentesse, e in particolare quelli che provengono da famiglie più deboli, di avere un percorso sostenibile. Questo provvedimento allontana tutto questo,

economicamente e socialmente più svantaggiati. Poi c'è il terzo punto che è oggetto di questo emendamento, importante quanto gli altri: è il punto della qualità

che le università private telematiche non avrebbero avuto accesso ai corsi di formazione. Avete bocciato tutti i nostri emendamenti e addirittura bocciate adesso questo nostro emendamento che cita i requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale. Colleghi, non si può giocare sul tema della qualità nel nostro sistema universitario!

le condizioni studentesche, anche sul tema della qualità, dice quanto questo vostro provvedimento, che sbandierate come un passaggio decisivo, in realtà sia un contraccolpo molto pericoloso.

impegna il Governo a garantire un accesso programmato, progressivo e sostenibile al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, in coerenza con il fabbisogno del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale

intaccare questa realtà verticale, di *élite* estremamente chiusa (non a caso l'ossimoro parla di chiusura), si irritano, gridano al pericolo e addirittura evocano fantasmi di chissà quale realtà negativa. Ma siamo tutti folli? Penso proprio di sì. In certi momenti la politica, quando è incapace di recepire una realtà positiva, impazzisce. Noi psichiatri lungimiranti abbiamo

dette con un po' di difficoltà fisica, forse daranno fastidio a qualcuno. Vi è una specie di disconferma della realtà che porto avanti. Come direi al caro presidente Zaffini, dico pensieri che non condivido, ma in questo caso li condivido con coerenza con le mie parole. È assolutamente incredibile gridare allo scandalo se si dice, contemporaneamente che bisogna abolire il numero chiuso e, nel contempo, nulla avete fatto per abolirlo, anzi, ne avete timore. La verità è una.

nel 1964 decisi di iscrivermi al corso di medicina. Lo facevo per passione, per vocazione, ma anche per rabbia, perché il mio amato padre, il mio bisnonno,

Nacqui asfittico e venni rianimato, anche se, subito dopo la guerra, essere rianimato era un po' complesso.

Il numero chiuso non c'è. Il numero chiuso era dato dal mio rendimento all'università. Scelsi «La Sapienza» prima e la «Cattolica» per la specializzazione in neuropsichiatria. Ero condannato a voti alti, detto: questo con disabilità - mi pare che ero il secondo in Italia - che ha avuto il vizio di vivere e vuol fare questa carriera così complessa, se non è almeno bravo vuol dire che sarà scadente sia a livello psicofisico che cognitivo. Negli anni tentai di dimostrare che forse, come i miei parenti quando assistettero al parto di mia madre Leonilde, avevano sbagliato. Sono giunto, senza nessun narcisismo, a anche l'istituto italiano di salute pubblica più antico, ossia l'Istituto italiano di medicina sociale, e devo dire che non mi sono vendicato mai con nessuno, se non con proposte indecentemente logiche. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi e colleghe, il numero chiuso non ci può e non ci deve essere, ma la colpa è di chi l'ha mantenuto per troppo tempo. Non ci sono scuse.

potuto vivere migliaia di persone, potenzialmente studentesse e studenti di una facoltà di medicina chiusa, come poteva esserlo per me; per fortuna in anni antichi non era chiusa, se non forse dal pregiudizio

forse c'è poca rabbia; non la rabbia violenta che crea le guerre, dalla famiglia al quartiere, al paese contro paese, la rabbia di voler cambiare le cose, come dicevo oggi nel mio ufficio, con grande dolcezza.

se lo facevamo noi - e non l'avete fatto - era cosa buona e giusta; se lo fa la maggioranza con coraggio, con forza, con complessità, pare che tutto sia sbagliato. Colleghe e colleghi, sinceramente non voglio fare il grillo parlante, anche se sono un esperto di Pinocchio.

colleghe e colleghi, prima di tutto voglio ringraziare il relatore e presidente della 10a Commissione Zaffini, il presidente Marti e tutte le colleghe e i colleghi delle due Commissioni competenti 7a e 10a,

purtroppo - e sottolineo purtroppo - voterà contro questo provvedimento e spiegherò i motivi che ci hanno indotto a questo voto contrario. dire in premessa alla Sottosegretaria, che ringrazio sempre per la disponibilità che ha dimostrato nel corso del lavoro delle Commissioni riunite e durante le audizioni, che noi siamo noi siamo e rimaniamo favorevoli all'abolizione dell'attuale *test* di ingresso per la facoltà di medicina,

Questo è un punto che voglio mettere subito agli atti in questa dichiarazione di voto del Gruppo Italia Viva. Su questo punto siamo assolutamente d'accordo

con grande delusione delle famiglie e degli studenti, che hanno investito risorse molto importanti e hanno perso mesi e mesi di studio e non solo di tempo, da questo punto di vista. Ma, proprio per queste ragioni, noi non abbiamo compreso perché allora non si è cercato di fare un provvedimento strutturale,

un euro in più. *(Applausi)*. Questo - mi dispiace dirlo - è l'ennesimo manifesto di propaganda, che va bene per i titoli dei giornali del giorno dopo («Abbiamo abolito il numero chiuso»), sapendo che il numero chiuso - l'avete detto anche voi - non lo si va ad abolire, ma soprattutto non si va ad incidere sui veri cambiamenti che abbiamo la necessità di adottare per colmare le odierne macroscopiche diseguaglianze sociali (che ci sono già adesso, proprio per le ingenti risorse che le famiglie devono spendere). Andiamo addirittura a peggiorare le diseguaglianze che già oggi sono in atto: per la serie, se se hai poche risorse, sicuramente avrai meno possibilità di continuare a frequentare la facoltà di medicina, deprimendo ancor di più la possibilità di far emergere i talenti, i migliori che noi abbiamo e che dovremmo continuare a selezionare, aumentando e potenziando la qualità formativa, non abbassandola. Questo è uno dei motivi che ci spinge e che ci ha spinto ad andare verso il voto contrario. Avremmo voluto, in questo caso, parlare di programmazione, come è stato detto in tutti gli interventi, anche nella discussione generale di ieri, di potenziamento delle aule universitarie e dei laboratori. Se si conosce la realtà delle università, sappiamo già dai numeri che abbiamo oggi - ed è stato spiegato anche ieri - che le facoltà, così come sono strutturate,

i medici vanno pagati di più. *(Applausi)*. Vanno assunti nuovi medici, certamente, ma dobbiamo recuperare un rapporto di fiducia tra medico e paziente che oggi si è perso e fare in modo che anche le altre specializzazioni abbiano la stessa empatia

ai patologi. Abbiamo bisogno di investire in tutte le specializzazioni e sappiamo quanto lo Stato investe nella formazione

circa un miliardo e mezzo. Abbiamo la necessità di aumentare la qualità formativa e quindi la qualità dei nostri studenti che si andranno a laureare e specializzare. Dobbiamo evitare, invece

È il motivo per cui se, da una parte, parliamo di carenza del personale medico, con tutte le cose che ho detto prima, dobbiamo poi capire, dall'altra, come programmare i numeri per i prossimi anni, sapendo che tanti medici andranno in pensione.

contrario? Oggi non scrivete in maniera chiara che la qualità formativa e didattica andrà a diminuire (perché oggi non è scritto che si apre alle università private telematiche) ma si dà una delega in bianco al Governo, cioè dopo che le Commissioni parlamentari hanno lavorato e dopo aver presentato cinque disegni di legge, si decide che dopo il primo semestre, lasciamo il caos. Non diciamo agli studenti che si iscriveranno il prossimo anno cosa succederà. Diamo infatti una delega in bianco al Governo che, senza mettere una risorsa in più, dovrà decidere quale sarà il destino

che stimo moltissimo e lei lo sa, perché non abbiamo pensato di fare una riforma strutturale, approfittando di questo momento, prendendo anche più tempo, ma cercando di fare

a quello che sta venendo fuori dalla manovra finanziaria, c'è una scelta ben precisa, c'è una direzione di questo Governo, indipendentemente da alcuni decreti-legge e provvedimenti, su cui, quando sono positivi,

Ecco perché - vi è stato detto anche durante le audizioni - noi saremo sempre al vostro fianco quando varerete provvedimenti che vanno nella direzione di migliorare la qualità della vita e soprattutto la qualità del futuro dei nostri giovani. Purtroppo, non escludendo in maniera definitiva la possibilità di aprire anche alle università telematiche, pensiamo che ci sarà ancora una volta un terreno di scontro ideologico, in cui forse solo alcuni si avvantaggeranno

Guardando, infatti, alle università telematiche in particolare, come possiamo pensare che uno studente in medicina possa fare pratica, ad esempio, nei laboratori? Ricordate il gioco del piccolo chirurgo con i pulsantini? Ecco, mi sembra di vedere la stessa cosa. I ragazzi devono fare pratica, gli studenti devono andare nei laboratori, devono fare e toccare con mano quello che sta succedendo e avere docenti

nella discussione generale di ieri, che siamo di fronte ad un provvedimento che, almeno secondo noi, in questo caso non è soltanto propagandistico ma è un vero e proprio provvedimento ingannevole da parte di questo Governo. Sì, perché nonostante sia stata fatta in queste settimane una vera e propria campagna mediatica in merito alla cosiddetta abolizione del numero chiuso per il corso di laurea in medicina e in chirurgia,

illusioni che penso sarebbero molto sbagliate tra gli studenti e tra le famiglie. La cosa che si fa è spostare la cosiddetta tagliola a sei mesi dopo, con tre materie - fisica medica, biologia cellulare genetica e i princìpi di anatomia umana - comuni tra i corsi di medicina, biotecnologie mediche e scienze motorie e sportive a cui si accede liberamente, ma solo coloro che avranno superato i tre esami previsti potranno poi continuare il percorso ed eventualmente - ma questo lo vedremo nei prossimi mesi - partecipare ad un ulteriore test nazionale per proseguire nel corso di laurea in medicina. Tutti gli altri, quelli che non riusciranno a passare questi tre esami e un eventuale nuovo test, potranno soltanto continuare gli studi in biotecnologie mediche o in scienze motorie o iscriversi ad un altro corso di laurea. In altri termini - altrimenti, veramente chi ci ascolta fa fatica a comprendere fino in fondo - quello che succede è che si sposta di sei mesi la selezione per coloro che invece vorrebbero effettivamente frequentare la facoltà di medicina, determinando un meccanismo che, a nostro avviso, peserà in termini di impegno e di costi economici, addirittura più di quanto accada oggi. Del resto, si è avuta pochi minuti fa la prova del nove di quello che sto dicendo: la mia forza politica, Alleanza Verdi e Sinistra, che da sempre si batte contro il numero chiuso, ha presentato un solo emendamento a questo provvedimento, emendamento - quello sì

Qui non si sta né superando il numero chiuso, né superando il test di ingresso, che viene soltanto spostato più avanti. Peraltro, il sistema delle barriere d'accesso, delle alte tasse e del numero chiuso ha ridotto la qualità della formazione e il numero delle persone laureate. L'università attuale non è più uno strumento per migliorare la condizione sociale delle persone, anzi, purtroppo è profondamente segnata da una dimensione classista; lo stesso accesso ai gradi superiori della formazione, come sappiamo, è un percorso ad ostacoli: dottorati senza borse, contratti a salari zero, corsi di formazione postlaurea spesso inutili, dipendenza mortificante dall'ordinario, un totale scollegamento con il mondo del lavoro. All'inizio del ciclo delle riforme,

a un processo di dequalificazione, di scarsa valorizzazione delle capacità di chi entra nel sistema della formazione. Purtroppo siamo l'unico Paese nel mondo industrializzato che non considera il finanziamento alla formazione pubblica per quello che è, cioè uno strumento anticiclico, esattamente inteso come un modo per contrastare la crisi, per frenare gli effetti nefasti della precarizzazione, per esempio, del mondo del lavoro. Ebbene, noi crediamo da sempre che il numero chiuso sia uno strumento sbagliato, ingiusto, inaccettabile; che le università non riescano a fornire i servizi che dovrebbero, perché non sanno garantire il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. Questo succede perché le risorse dello Stato L'attuale modello a numero chiuso è profondamente penalizzante, soprattutto per quegli studenti che provengono da contesti familiari e sociali più disagiati, da territori più marginalizzati. La necessità di sostenere dei costosissimi corsi preparatori ai test d'ingresso crea una barriera davvero socioeconomica nei confronti delle persone più deboli. Come ben si vede, il problema non è, quindi, soltanto nel numero chiuso o nei test, ma nella mancanza di investimenti strutturali nel sistema universitario pubblico e naturalmente anche, in questo caso, nella sanità pubblica. Senza risorse aggiuntive per migliorare le infrastrutture, per ampliare i corsi, per aumentare il personale, l'abolizione del numero chiuso risulta una promessa vuota, che non affronta le vere necessità del settore e, come purtroppo accade da troppi anni a questa parte, invece di investire maggiormente nell'istruzione, nell'educazione, lo Stato risolve tagliando il numero degli aventi diritto. Qualche mese fa,

di docenti, di ricercatori e di personale, quindi di fatto ridurre la possibilità di accesso al diritto allo studio pubblico. Di contro - e su questo davvero esprimiamo un grande dissenso - semplificate le norme per le università telematiche,

quello del presunto superamento del test d'ingresso, di fronte a un sistema che produrrebbe l'espulsione di oltre 40.000 studenti ogni anno, naturalmente con un sovraffollamento nel primo semestre, che non so bene come si pensa di risolvere senza soldi e senza investimento; forse con i corsi da remoto, perché non vedo un altro tipo di soluzione. Davvero non si capisce come tutto questo possa essere sostenibile senza un incremento del fondo di finanziamento ordinario. Noi abbiamo voluto presentare quel solo emendamento esattamente per dimostrare come davvero in questo caso siamo dinanzi a una operazione molto poco concreta, molto propagandistica, che non metterà le università nella reale condizione di accogliere studenti e studentesse senza abbassare la qualità. Per tutte queste ragioni che ho detto, come Alleanza Verdi e Sinistra siamo contrari al provvedimento in esame. Vi chiediamo, invece, ma non da oggi, da sempre, di garantire la salvaguardia del sistema pubblico che state purtroppo contribuendo a smantellare. Il numero chiuso, dal nostro punto di vista, lo dico ancora una volta, rappresenta davvero una barriera sociale e culturale che pensiamo vada superata, ma che si supera soltanto attraverso provvedimenti che prevedano risorse. Non servono misure *spot*, non serve illudere gli studenti, non serve illudere le famiglie, serve investire nell'università pubblica e nella sanità pubblica. Servono più medici, com'è stato giustamente detto ieri più volte, anche perché - come sappiamo - le strutture di pronto soccorso esplodono, il personale sanitario deve fronteggiare ogni giorno un'emergenza continua ed è spesso sottoposto ad orari di lavoro e turni massacranti. Servono insomma reali e concrete risposte in un Paese nel quale ormai - lo sappiamo bene e davvero questo dato deve interrogarci profondamente - quasi 5 milioni di persone hanno hanno smesso di curarsi. Allora - ho finito davvero - servono risorse, servono provvedimenti strutturali; altro che gli astratti riferimenti al merito, altro che sviluppare ancora di più come avverrà inevitabilmente - una competizione tra gli studenti che all'interno del sistema universitario - io credo - non dovrebbe esistere. Per tutte queste ragioni, come Alleanza Verdi e Sinistra voteremo contro questo provvedimento. Signor Presidente, ci tenevo a svolgere questo intervento perché quello di oggi è un traguardo molto importante, perché noi volevamo che si arrivasse a questa tappa che ha visto molto impegnata il ministro Bernini e tutto il Governo proprio per l'abolizione di questo meccanismo un po' infernale dei quiz. Vedete, l'uomo politico che vive a contatto con la realtà ascolta cittadini, persone che rappresentano istanze. In tutti questi anni ho toccato con mano la disperazione di genitori che hanno spedito questi ragazzi un giorno a Roma, un giorno a Napoli, un giorno a Pavia, poi siamo arrivati alla ex Jugoslavia che ha creato nuovi Stati, con facoltà universitarie. Poi abbiamo università italiane, anche romane, che hanno delle diramazioni in Albania. Quindi ho seguito l'evoluzione del tema ascoltando la gente, perché un politico che vive la vita quotidiana parla col generale, parla con il fioraio, parla col contadino e parla con la famiglia alle prese con un'aspirazione. Dopo di che noi abbiamo un problema, uguale e contrario: la mancanza di medici. Per cui dobbiamo prendere medici e infermieri dall'estero. Poi capisco che c'è anche un problema di pagamenti, di trattamenti economici e quindi la galassia della medicina è molto problematica. Vede, ministro Bernini e Sottosegretario, anche quest'anno che abbiamo stanziato - voi come Governo - la cifra record di circa 136,5 miliardi (cito a memoria, miliardo più, miliardo meno), c'è chi si lamenta, dimenticandosi a sinistra dei tagli che hanno realizzato.

Però poi vedo che il fondo del finanziamento ordinario - chiedo che anche questo resti agli atti, lei ne ha parlato anche ieri - è più alto rispetto all'anno precedente: tocca 9,2 miliardi nel 2023, 9,04 nel 2024 e 9,21 nel 2025. Poi ci sono i finanziamenti per i laboratori, in base alla legge n.

per finanziare nuove infrastrutture. Vi siete occupati degli studentati (io faccio parte di una generazione che li chiamava «la casa dello studente», ma ho scoperto che si chiamano studentati, che non mi piace molto, però chiamiamoli così): però chiamiamoli così): quindi l'accoglienza, la residenza degli studenti, i fuorisede. Quindi, anche l'accesso a medicina credo che lo abbiate realizzato con una fase di ascolto, con valutazioni condivise e anche con la mediazione delle forze politiche. Non so sul voto finale, ma mi auguro che tutti si uniscano a questo traguardo e chi non si unisce fa male. Oggi hanno detto quelli dell'opposizione che il Governo e la maggioranza sono divisi. Nell'arco di trentasei ore noi variamo al Senato un provvedimento fondamentale per l'accesso alle facoltà di medicina, che interessa le famiglie, la sanità, gli studenti e la medicina del futuro. Quando in questi giorni mi chiedevano che pensavo del canone della Rai, dicevo ai giornalisti che mi stavo occupando dell'accesso alle facoltà di medicina, perché è un tema socialmente più importante per chi ci vuole entrare e per chi vuole essere curato. Invece tutti devono parlare di argomenti che, lo capisco, sono politicamente più divertenti, ma per cento di noi: i cinquanta giornalisti che ci fanno la domanda e i cinquanta tra noi che hanno la fortuna di essere chiamati a rispondere. Noi oggi approviamo questo testo come maggioranza unita. Mi sembra Camera abbiano concluso o stiano concludendo il decreto sui flussi. Una vicenda complicata, con l'immigrazione, l'Albania, i Paesi pericolosi e quelli sicuri, e il Governo l'ha affrontata.

le modalità di questo test unico nazionale, introdurrà un modello originale, con un programma di studi comune che consentirà poi ad uno studente meritevole di essere indirizzato verso un percorso formativo. Non vogliamo abolire i quiz perché vogliamo che tutti facciano i medici. Tutti noi vogliamo essere curati da professionisti competenti quando avranno concluso il corso di studi, ma vogliamo che sia il corso di studi a verificare le qualità, gli orientamenti, le attitudini e a dire ad uno studente: se non ce la fai, se non sei adatto, fai altro. Questo perché un medico in mano la vita di tutti quanti noi.

è un problema parallelo. Ci è stata rivolta una critica: l'accesso e i quiz non sono la soluzione al numero chiuso. State lavorando anche su questo, valutando l'autonomia dell'università, valutando tutte le competenze, la CRUI e i rettori, che rispettiamo. Io non voglio essere iconoclasta. Noi vogliamo

essere più generosi anche con l'azione del Governo. Saranno i crediti formativi a regolare l'accesso e la posizione raggiunta in una graduatoria nazionale. Vi sarà un orientamento dalla scuola secondaria, che è fondamentale. Signor

perché è nella sua tradizione familiare. Io poi credo a queste cose, perché avere degli studi alle spalle, avere avuto dei buoni insegnamenti, non è indispensabile: ciascuno può, nella scala sociale, partire dal punto più lontano ed arrivare al punto migliore. Ma per lei, che ha una tradizione a cui è molto legata e a cui tiene, credo che realizzare questa riforma, che è solo una parte delle tante altre cose che sta facendo, sia una particolare soddisfazione. Mi avvio alla conclusione, orgoglioso, come Gruppo Forza Italia, questo consentitemelo, di approvare questo provvedimento. Era una delle misure di cui anche col presidente Berlusconi si discuteva. A volte ci si interrogava dicendo: come mai mancano i medici? Ci sono questi quiz assurdi. Non si può creare un meccanismo che verifichi le capacità e le attitudini?

sarebbero chiusi gli ospedali e le corsie. Abbiamo tanti giovani capaci e volenterosi. Quindi, non si affidi più questa selezione a una specie di terno al lotto. I quiz lasciamoli agli spettacoli serali della televisione, dove uno va, risponde, prende un sacco di soldi;

Allora, se c'è un test che deve valutare chi può fare il medico e chi no, dovrebbe tener conto di questo, ossia della predisposizione a svolgere quella missione. L'attuale test è invece quello che tanti colleghi hanno definito - e io condivido - ingiusto, iniquo, in realtà inaccessibile soprattutto a quei ragazzi che provengono da famiglie economicamente più svantaggiate. L'essere diventato così iniquo e così ingiusto in realtà è accaduto anche un po' nel tempo. Sono una dei medici che è entrata a medicina con il numero chiuso, e credo fosse uno dei primi anni in cui fu introdotto il numero chiuso. Eppure all'epoca, senza aver fatto alcun corso privato, anche perché provenivo da una famiglia economicamente umile, mi preparai da sola utilizzando i libri di testo e riuscii ad entrare. Nel tempo, però, la preparazione a quel test è diventata un vero e proprio mercimonio: abbiamo visto il pullulare di test e di corsi privati che approfittavano della debolezza, della fragilità, anche della disperazione delle famiglie, soprattutto di famiglie in difficoltà, per fare profitto. E questo è vergognoso. Signor Ministro, come lei, conosco tante storie di ragazzi che avrebbero voluto fare il medico e non l'hanno fatto, perché hanno dovuto rinunciare a quel sogno. Penso a Rosa, che sarebbe stata un brillante medico e che voleva andare a lavorare nei teatri di guerra e nei Paesi poveri, ma oggi fa un dottorato in Argentina non per fare il medico, ma per fare altro, perché a quel sogno ha rinunciato per pochissimi millesimi di punto. Penso a Ciro, che ha fatto il test di ammissione a medicina qualche mese dopo aver perso il padre per un tumore, e forse provare a fare il medico era anche in qualche modo un voler onorare la memoria del padre. Un po' come è stato per me scegliere di fare medicina dopo la morte di mio nonno: anche io io all'epoca volevo trovare la cura contro il cancro. Signor Ministro, quando si rinuncia a un sogno, quando si rinuncia a svolgere una missione per cui ci si sente portati, penso che in realtà nel cuore resti sempre quel sogno che non viene mai dimenticato. E poi c'è un altro fattore di cui nessuno ha parlato finora. In realtà, qualsiasi cosa alternativa si scelga di fare, l'ingresso a un'altra facoltà o un altro lavoro, è come se partisse già su un fallimento. Noi abbiamo condannato per anni dei giovani a rinunciare al sogno e ad accontentarsi di qualcosa che magari non era la loro aspirazione principale. Per non parlare poi di chi ha avuto invece la possibilità economica di fare ricorso al TAR e poi è entrato a medicina, o di chi - come lei ricordava, signor Ministro - ha avuto la possibilità economica di frequentare l'università all'estero, il cosiddetto esilio universitario. Davvero in questi anni purtroppo l'accesso a medicina è stato non meritocratico, non ha valorizzato le aspirazioni e le vocazioni C'è un altro punto. Noi in quest'Aula, soprattutto, dobbiamo parlare sempre di più di come garantire a tutti i cittadini i diritti sanciti nella nostra Costituzione, e diritti ce ne sono almeno due in questa legge. in questa legge. C'è il diritto allo studio, sancito dall'articolo 34 della Costituzione, che dice che tutti i ragazzi meritevoli, anche se appartenenti a famiglie economicamente disagiate e anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Poi c'è l'articolo 3, che dice che lo Stato deve eliminare qualsiasi ostacolo che impedisca la piena realizzazione della persona umana. Realizzare il proprio sogno, mettere a frutto il proprio talento, realizzare la propria vocazione significa proprio questo: permettere alla propria persona di svilupparsi. *(Applausi)*. Per tutti questi motivi, Ministro,

perché convinti che questo fosse un tema a cui doveva lavorare tutto il Parlamento, in maniera trasversale, proprio per garantire quei diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Devo dire che in questo testo unificato rivedo tante delle nostre proposte e rivedo tanto di noi, e l'ho ricordato prima, mentre discutevamo gli emendamenti. Eravamo partiti con due canali separati: da un lato, la provenienza dal liceo biomedico e, dall'altro, il semestre comune. Poi invece il canale biomedico è stato separato e incluso come crediti formativi aggiunti. Rivedo per esempio l'aver mantenuto la programmazione pre e postlaurea, che per noi era un punto fondamentale, inserito nel testo grazie all'apporto del MoVimento 5 Stelle. Ringrazio lei, Ministro, la Sottosegretaria, il relatore Zaffini, il presidente Marti e tutti i colleghi della Commissione, di maggioranza e di opposizione, perché credo che abbiamo fatto veramente un buon lavoro. Perché è importante questa programmazione? Ho sentito raccontare ed elencare numeri che non corrispondono sempre alla realtà. Quello che è mancato, da un decennio a questa parte, è stata proprio una corretta programmazione dei medici in base al fabbisogno di salute della popolazione. Sa perché? Addirittura fino al 2018, quando noi siamo arrivati al Governo, non c'erano posti di specializzazione a sufficienza per tutti i medici neolaureati. Cioè fino al 2018 avevamo 6.000 posti di specializzazione, a fronte di 10.000 laureati; quindi, si era creato un imbuto formativo per cui i medici si laureavano, ma non tutti potevano specializzarsi. E un medico senza specializzazione non può lavorare in ospedale. Fortunatamente, grazie ai nostri Governi, quell'imbuto formativo è stato colmato, perché oggi i posti di specializzazione sono oltre 13.000 e, quindi, anche la programmazione è migliorata. Le previsioni dicono che oggi abbiamo più o meno 100.000 medici ospedalieri; nei prossimi cinque anni 30.000 di questi andranno in pensione, però ce ne sono 60.000 già in formazione. Quindi, per il 2027 quel saldo negativo verrà però, è fondamentale programmare quali sono gli specialisti che ci serviranno. È chiaro che, non facendo figli, non ci servono tanti ginecologi, ma ci servono invece tanti medici di cure primarie per rafforzare il territorio; ci servono internisti, medici di pronto soccorso, di cui c'è una grave carenza. Ministro, ancora una volta le chiedo di ripensare a quel provvedimento che ha abolito quella tecnostruttura, che invece era utile e serviva a mettere in comunicazione l'Osservatorio scuole di specializzazione con l'Agenas, proprio per la programmazione. Un altro punto importante che rivedo nel disegno di legge e che noi abbiamo voluto inserire è la graduatoria unica nazionale e il fatto che i test previsti alla fine di questo primo semestre debbano essere *standard*, uniformi su tutto il territorio nazionale, per evitare che ci siano disparità nel Paese e anche disparità da docente a docente. Avevamo chiesto di fare attenzione anche a un'altra cosa, che è stata approvata in Commissione come ordine del giorno e che spero poi entri nella delega:

Purtroppo però, Ministro, nonostante abbia visto quanto io sia convinta che abbiamo fatto fino alla fine un buon lavoro, restano delle criticità. E questo è il motivo per cui alla fine noi ci asterremo sul provvedimento. Le criticità sono soprattutto due: la prima, le risorse. Lei ha detto, anche nella replica di ieri, che è evidente che serviranno delle risorse; per aggiungere solo 13.000 posti, quest'anno sono serviti 23 milioni di euro. Noi ci aspettiamo che, pur non avendo inserito nella delega la previsione di impegno di spesa, quando essa verrà sviluppata, verranno

pur non essendo le università telematiche accreditate per i corsi di medicina, dovendo fare un semestre comune a più corsi di studio, che poi il Ministero deciderà quali sono (farmacia, biotecnologia, biologia), ci sono delle università telematiche che hanno questi accreditamenti. A nostro avviso, quindi, serve mettere un paletto proprio per evitare che, avendo fatto uscire dalla porta quelle università, poi esse rientrino dalla finestra. finestra. L'astensione è anche motivata dal fatto che c'è un altro passaggio alla Camera in cui speriamo che questi correttivi vengano

continuare a lavorare anche alla formazione post laurea. Sono felice che proprio in queste settimane in 7a Commissione si stiano discutendo altri due provvedimenti importantissimi che sempre lei, Ministro, ha voluto inserire all'ordine del giorno: uno relativo alla formazione specialistica dei medici e l'altro sul pre-ruolo dei ricercatori. Anche su questi provvedimenti ci vedrà impegnati sempre in maniera costruttiva, come siamo abituati a fare. Serve però un impegno importante per valorizzare sempre di più i medici in Italia. Oggi un medico ospedaliero viene pagato 80.000 euro a fronte dei 150.000 di un medico tedesco. È chiaro che, se non paghiamo meglio questi medici, se non mettiamo un argine ai gettonisti, cioè a quei medici che, pur non essendo dipendenti del Servizio sanitario nazionale, lo aiutano facendo turni molto più leggeri e guadagnando tre volte tanto, noi continueremo a perdere personale e non ce lo possiamo permettere. Tutto questo, Ministro, solo per dirle che, ogni volta che lei farà una battaglia a difesa dell'università e del diritto allo studio, ci troverà sempre al suo fianco. Le voglio però anche dire

poiché durante i lavori parlamentari in cui è in discussione la legge di bilancio è previsto un taglio ai Ministeri e anche al Ministero dell'università e della ricerca, il finanziamento disponibile per la realizzazione delle iniziative finanziate, a valere sull'avviso piano nazionale complementare a titolarità ministeriale, risulta ridimensionato nei seguenti termini. Il ridimensionamento previsto in legge di bilancio, se confermato, determinerà la necessità di una rimodulazione di questi che sono progetti di ricerca già finanziati e, poi, si dice anche che la scrivente amministrazione ha presentato proposte emendative volte al recupero parziale dei menzionati abbattimenti. Vede, Ministro, lei non deve presentare emendamenti. Noi, come opposizione, dobbiamo presentare emendamenti. Lei, come Ministro e voi, come maggioranza, dovete mettere al centro dell'agenda politica gli investimenti e sull'università, sul diritto allo studio, sulla ricerca e lo sviluppo. È infatti questo il settore che ha il più alto fattore di rendimento. Anche nei momenti di difficoltà in questi settori, Ministro, non bisogna mai smettere di investire. Se lei fa questa battaglia, le prometto che noi saremo al suo fianco. Signor Presidente, colleghi, Ministro, oggi assistiamo alla prima tappa di una rivoluzione che gli studenti italiani aspettano da appena Quella che arriva all'esame dell'Assemblea oggi, dopo una gestazione lunga e meticolosa della Commissione che mi onoro di presiedere, è una riforma ambiziosa che intende potenziare il Servizio sanitario nazionale in termini sia di numero di medici chirurghi, sia di qualità della loro formazione. Abbiamo ascoltato davvero tutte le parti in causa:

facendo tesoro del contributo - anche critico - offerto. Abbiamo parlato con i medici, con gli specializzandi, con le tante società private che fino ad oggi hanno lucrato sulla preparazione ai fantomatici test e abbiamo anche ascoltato gli studenti, che ci hanno chiesto di trovare un sistema capace di dare valore al loro studio e al loro sacrificio. Abbiamo lavorato in un comitato ristretto partecipatissimo, in cui tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione si sono messe in gioco per superare ognuno la propria idea e permettere l'approdo a un risultato il più possibile condiviso e ottimale per il Paese. Mi permetto di ringraziare il ministro Annamaria Bernini, tutti i suoi uffici e Massimo Rubechi per il costante il relatore, Francesco Zaffini, che non solo è il relatore, ma è anche il Presidente della 10a Commissione (sanità) e che in modo un po' irrituale ho voluto che svolgesse questo ruolo su un provvedimento assegnato come competenza alla 7a Commissione,

lo si sia svolto tutti insieme, scegliendo la soluzione migliore, che è quella di tenere unito il mondo dell'università, con il Ministro presente, la Presidenza della Commissione affari sociali e sanità e chiaramente coinvolgendo - come è giusto che sia - anche il Ministero della pubblica istruzione e del merito. Ringrazio, rigorosamente in ordine alfabetico, le senatrici Aloisio, Bucalo, Castellone e D'Elia e i senatori Crisanti, Occhiuto e Paganella, che hanno lavorato insieme a noi al comitato ristretto il mio ringraziamento va quindi a tutti voi per il lavoro svolto. La stella polare che abbiamo avuto in questo lavoro è stata la nostra Costituzione. Quando il Governo eserciterà la delega che gli stiamo conferendo, finalmente si darà attuazione al diritto alla salute - da un lato - a quello all'istruzione - dall'altro lato - sempre nel pieno rispetto dell'autonomia dell'università. In ragione della complessità della materia, la formazione dei medici, ovvero il futuro globale del nostro Paese, abbiamo scelto di optare per la legge delega. Già come primo firmatario, avevo previsto un ora il Ministro dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero della salute, dell'istruzione e del merito e quello delle finanze con la conferenza Stato-Regioni, ha dodici mesi per emanare i decreti legislativi che diano attuazione ai principi che abbiamo enucleato. L'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea finalmente sarà libera: non esisterà più il test di accesso. Il semestre diventa dunque un filtro, un periodo di sei mesi e non più di un paio di ore come nel sistema attuale che da venticinque anni svilisce i giovani e genera un'enorme mole di contenzioso, in cui i ragazzi avranno così modo di dimostrare le loro vere capacità e le competenze acquisite con la frequenza dei corsi e con lo studio individuale.

Si tratta, quindi, di riordinare complessivamente l'offerta formativa di tutta quest'area universitaria, a partire dall'allineamento dei corsi del primo semestre. Al momento dell'iscrizione al primo semestre, ciascuno studente si iscrive gratuitamente anche ad un secondo corso di studi della medesima area, che costituisce così la sua seconda scelta. Gli esami di profitto di queste materie saranno svolti secondo degli *standard* uniformi e su questo voglio essere ancora più chiaro: non ci sarà alcuno spazio per scorciatoie e favoritismi, come abbiamo più volte sottolineato e come il Ministro ha garantito. in una università piuttosto che in un'altra non potrà in alcun modo dare un vantaggio o, viceversa, uno svantaggio. Si garantirà assoluta parità di condizione tra tutti gli studenti. Gli studenti che abbiano superato tutti gli esami del primo semestre entreranno in una graduatoria di merito, che potrà garantire l'accesso al secondo semestre di medicina, odontoiatria e veterinaria. Coloro che non si saranno collocati in posizione utile per accedere a medicina, odontoiatria e veterinaria potranno proseguire il secondo semestre nel corso di studi di seconda scelta, anche in sovrannumero. Questo non è banale: la specifica «anche in sovrannumero» è stata introdotta con un emendamento a nostra prima firma, dal momento che la maggior parte dei corsi di studio di area biomedica - come sappiamo tutti - prevede il cosiddetto numero chiuso di ateneo, cioè offre un numero limitato di posti. Si riconosce e si tutela così il valore di ciascuno studente. Chi, invece, non avrà completato gli esami del primo semestre potrà proseguire gli studi nel corso di seconda scelta, se ad accesso libero, oppure iscriversi tardivamente a qualsiasi altro corso di studi. Nessuno, quindi, perderà tempo o si vedrà schiacciato da un sistema ingiusto. In ogni caso, l'anno successivo chi lo desidera potrà iscriversi nuovamente al primo semestre libero e avere una nuova *chance* per proseguire gli studi in questi corsi. Lasciatemi dire qual è la grande portata del disegno di legge in esame: si prevede il potenziamento della programmazione annuale del numero di accessi alle facoltà di medicina, odontoiatria e veterinaria. Parliamo non di una maggiorazione di qualche manciata di posti, ma di misure strutturali e di modifica dei criteri di calcolo, ovvero di un effettivo superamento del meccanismo in uso, che ha mostrato tutti i suoi limiti, anche e soprattutto durante l'emergenza sanitaria. Il Governo dovrà anche potenziare la capacità ricettiva degli atenei, sempre continuando a garantire elevati *standard* di qualità dell'insegnamento. A tal proposito, un emendamento della Lega introduce la previsione di criteri di sostenibilità delle iscrizioni al primo semestre, rispetto alla capacità di accoglienza in ciascun ateneo. A mero titolo di esempio si potrà prevedere l'erogazione dei corsi puramente teorici a distanza, con modalità sincrone e asincrone, e si potranno prevedere criteri di bilanciamento tra gli atenei limitrofi. Per raggiungere questo obiettivo si prevede inoltre come noi abbiamo voluto fortemente - che le attività teoriche e pratiche dell'intero corso di studi in medicina e di tutoraggio degli studenti possano svolgersi anche in strutture sanitarie accreditate e negli istituti di ricovero e cura e carattere scientifico. Elemento importante

È così che si crea un primo filtro e si permette agli studenti di scegliere consapevolmente il percorso di studi più adatto. Sono davvero orgoglioso, colleghi, signora Ministro, che il disegno di legge in atto a mettere fine ai test di accesso a medicina: una battaglia che, come molti di noi, la Lega ha sempre portato avanti con determinazione da più legislature e che ora vede finalmente la luce, con l'auspicio che l'*iter* di questo provvedimento possa concludersi presto e nel migliore dei modi, per permetterci di archiviare quanto prima il fallimentare sistema attuale. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito

inviso a tutti. Qui si discute su un tema complesso, perché tocca un nodo strategico del Paese: il nesso tra qualità della formazione e qualità del diritto alla salute delle persone,

con l'idea di dare ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi che vogliono intraprendere questo percorso la possibilità di verificare la propria attitudine.

percorso lungo, perché non si è medici senza specializzazione. Quindi, anche solo affrontare l'accesso in modo isolato dal resto è fuorviante, perché il nodo è tenere insieme apertura ed eccellenza della formazione, che è cardine della qualità della cura delle cittadine e dei cittadini. Si ha la sensazione invece che qui abbiamo solo rimandato la soglia, senza aggredire davvero l'iniquità e neanche affrontare i temi reali di difficoltà. E lo dico avendo partecipato al percorso ed avendo sollevato alcune questioni di merito su quello che andavamo facendo. L'abbiamo detto: è iniquo il modo in cui oggi si accede. Cito Alessia Conte, tra i vari studenti che sono intervenuti in audizione, perché è la presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari, organismo che voi non volete tra gli enti che devono esprimere un parere su come si va a ridefinire, visto che avete bocciato il nostro emendamento. Ebbene, Alessia Conte ci ha fornito i dati su chi riesce ad accedere a medicina e poi ci ha anche voluto mandare tutto il rapporto Istat a dimostrare a tutti i membri della Commissione che al corso di medicina e chirurgia in questo Paese ancora oggi accedono studentesse e studenti con i redditi più elevati rispetto agli altri corsi. C'è una selezione che è fortemente ancora di classe. Quindi, ci sono due questioni: un'iniquità che nasce da una barriera in sé del sistema universitario, che per essere aperto a tutti dovrebbe garantire una didattica di qualità per quelli che vorrebbero fare questo percorso costoso e raggiungere poi un'iniquità che nasce dalla modalità in cui selezioniamo per ottenere un numero programmato che ci consenta di garantire quelle due qualità di cui parlavo. Ed è su questo che sono arrivati i rilievi critici: due piani, però, che in questa discussione si sono confusi più volte. Alcuni applaudono alla fine del numero chiuso che non c'è, illudono famiglie, ragazze e ragazzi con quella libertà di accesso che riguarda il semestre libero. Vorremmo evitare che sia una semplice dilazione, una bandierina da sventolare. Non si può cambiare accesso senza un percorso di adeguamento delle strutture di assunzione di personale, di potenziamento dell'orientamento in uscita dalle scuole: l'orientamento, non un anticipo di formazione universitaria *(Applausi)*, testo si dice. Anche qui, comunque, è tutto a invarianza finanziaria e più in generale è un investimento volto alla sostenibilità dell'apertura. Di cosa invece stiamo discutendo? Questo dobbiamo chiarirlo, perché già l'articolo 1 non corrisponde a verità. Le finalità dell'ampliamento, del potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di numero di medici, chirurghi, odontoiatri e veterinari non sono in questo testo. Qui c'è una delega per una revisione delle modalità di accesso. E quali sono i problemi da affrontare per allargare e potenziare davvero? Li possiamo prendere da due versanti: quello del Sistema sanitario nazionale parliamo dei problemi storici, della carenza di borse e di specialità rispetto al numero di laureati, un imbuto che in questi anni abbiamo affrontato, come veniva ricordato prima. La tendenza è stata invertita, ma mancano comunque di medicina generale e di medicina di urgenza. Poi c'è la questione dell'attrattività del Servizio sanitario nazionale: negli ultimi dieci anni 10.000 medici e 8.000 infermieri hanno lasciato per andare all'estero, dove sono pagati meglio, perché sono riconosciuti e il motivo è tutto economico. La media di un medico specialista in Italia è di 105.000 euro, mentre per i tedeschi e gli olandesi è di 190.000 e per gli spagnoli 108.000. Quindi, dove dobbiamo andare a guardare per capire se veramente finanziamo? Negli investimenti in università, ricerca e in quelli sul servizio sanitario nazionale. Ma gli investimenti non ci sono. In questa legge di bilancio non ci sono. Troviamo tagli nella dotazione del fondo nazionale in rapporto al PIL, che sarà al livello più basso. L'aumento di 1,3 miliardi è inadeguato a pareggiare l'inflazione e non c'è nulla per l'assunzione di medici e infermieri. Non si vede prospettiva da questo punto di vista, anche se è evidente che noi oggi ragioniamo di quello che sarà tra dieci anni. Ma allora vediamolo dal lato dei tagli sulla ricerca e l'università o degli investimenti sulla ricerca e università. Io non ho alcun pregiudizio, però vorrei parlare del *casus belli* di cui ieri abbiamo discusso, perché nasce dal parere espresso dalla CRUI sullo schema di riparto del fondo di finanziamento ordinario. Non è un comunicato

del fondo ordinario, perché ha un taglio contabile di 173 milioni di euro. Non risulta il finanziamento aggiuntivo di 340 della quota annuale del piano straordinario 2022, messo a carico del fondo ordinario, che prevedeva le risorse aggiuntive per aumentare le facoltà assunzionali degli atenei. La quota 2024 doveva essere quella più significativa. Con questo siamo a 513 milioni di tagli effettivi. Poi c'è la mancata copertura dei maggiori oneri derivanti dall'adeguamento degli stipendi del personale, obbligo a carico degli atenei stabilito dal MEF; oltre 230 milioni di euro di tagli per l'adeguamento di stipendi. La somma fa circa 750 milioni di euro di tagli certificati, stimati oltre 800. Non sono numeri a caso: sono mancati finanziamenti che il senatore Verducci, non si è inventato. Potremmo continuare, perché nel decreto n. 71 del 2024, avete tagliato altri 100 milioni alla copertura degli aumenti stipendiali del personale. Adesso, nella legge di bilancio c'è il blocco del *turnover* al 75 per cento rispetto alle cessazioni di ruolo e quel 25 cento di risparmio non andrà agli atenei e agli enti di ricerca, ma dovrà essere dato al MEF. Quindi, anche qui una stretta terribile. Così come ci sono i tagli sulle tabelle: alla ricerca, meno 366 milioni; alle università, meno 284; alle AFAM meno 50,4. Sono 122 le società scientifiche che hanno aderito all'appello di cui prima parlava la senatrice. C'è un tema serio di sostenibilità della ricerca e del futuro del sistema universitario, perché i piccoli atenei rischiano di fallire. E non possiamo discutere di questo, se non parliamo anche del contesto in cui noi mettiamo quella iscrizione libera al primo semestre. Questo è il cuore, che rischia di essere un enorme *bluff*. Questo semestre, infatti, come si organizza? Come risponde alla necessità di verificare la vocazione di queste ragazze e questi ragazzi? Io, che ho partecipato al comitato ristretto, non ho ancora capito come volete costruire questa graduatoria nazionale. E mi rifiuto di pensare che noi diamo dei crediti formativi universitari da remoto su test nazionali. Stiamo moltiplicando i test, solo che lo faremo, sulle materie di competenza. Stiamo cioè decidendo che un pezzo del percorso universitario sarà probabilmente fatto con i test a crocette e magari appaltato alle università telematiche. Su questo punto, infatti, non ci avete dato risposte ed è troppo facile scaricare sulle università telematiche e sull'insegnamento da remoto l'assenza di *welfare* e l'assenza di condizioni di qualità, per gli studenti e le studentesse, al fine di studiare nelle università. Per questo noi esprimiamo serie perplessità su questa legge delega, sulla vastità della delega, sul modo in cui si pensa di di fare la graduatoria e su cui si rischia di moltiplicare la competizione e lo stress, in sei mesi che non saranno sei veri mesi di verifica per i ragazzi e le ragazze. Per questo motivo, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.

questa sera sono orgogliosa di intervenire in dichiarazione di voto a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. Oggi stiamo infatti scrivendo una pagina importante per il futuro dei nostri giovani, garantendo a tutti la pari opportunità di diventare professionisti in ambito medico. Desidero innanzitutto ringraziare il ministro Bernini, che ha seguito e supportato costantemente i lavori nella 7a e 10a Commissioni riunite, il nostro relatore, il nostro relatore, il senatore e presidente Zaffini, e il presidente della 7a Commissione, senatore Marti, per il grande lavoro che è stato fatto con equilibrio e con efficacia per portare oggi in Aula questo disegno di legge. È stato un lavoro complesso, a partire dal raccordo di cinque disegni di legge, uno dei quali, il n. 915, di Fratelli d'Italia, a mia prima firma. Il testo è una legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. La riforma era attesa da anni, visto che l'attuale sistema basato sui test di ingresso a risposta multipla, come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, si è rivelato un sistema rigido, determinato da troppi fattori causali. Spesso il contenuto di alcune domande ha destato molte perplessità. ha mostrato sempre più la sua incapacità a selezionare con equità e merito gli studenti più bravi e motivati. Stiamo parlando del cosiddetto test lotteria. Il nuovo meccanismo parte invece da un assunto fondamentale: un sistema che permetta a tutti i ragazzi di avere il diritto di confrontarsi alla pari, di partire dagli stessi blocchi di partenza, al di là della scuola di provenienza, e di essere finalmente giudicati sul reale merito e sulle loro motivazioni. Inoltre, vale la pena dire a chiare lettere che abbiamo finalmente avuto il coraggio di eliminare il fiorire dei corsi privati che preparavano al *test* lotteria e che hanno notevolmente inciso sulle finanze di tutte quelle famiglie, che sono state costrette a pagare costi altissimi e che spesso hanno anche determinato un ingiusto divario per chi invece non poteva permetterselo. È prevista l'iscrizione libera a un semestre filtro: sei mesi di formazione in cui gli studenti si preparano su materie caratterizzanti e su cui verranno valutati secondo *standard* uniformi che saranno oggetto della delega. Il proseguimento al secondo semestre sarà regolato dal conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre e che saranno svolti in modo uniforme in tutti gli atenei. Smettetela quindi di dire che c'è il rischio serio di valutazioni non omogenee. La posizione utile in una graduatoria di merito nazionale, formata in base ai risultati raggiunti, seleziona poi l'ingresso al secondo semestre in base al numero dei posti programmati, il che garantirà la proporzione tra domanda e offerta. Sui criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre, basta con questi allarmismi lanciati anche da alcuni atenei secondo cui le strutture universitarie non riusciranno a garantire la capacità di accoglienza. Tutto ciò è assurdo e anacronistico. Siamo in una società sempre più digitalizzata, ci confrontiamo con l'intelligenza artificiale e voi venite a dirmi questo. Per alcune delle materie del primo semestre si potranno ampiamente utilizzare le tecnologie a distanza, visto che le abbiamo già utilizzate con successo nel periodo della pandemia e che sono state anche dalla CRUI durante la sua audizione. È stato previsto che gli studenti che non raggiungessero il posto nella graduatoria di merito utile a proseguire medicina

non perdono l'anno. Questa è la chiara e netta differenza con il modello francese, che in maniera del tutto falsa in questi giorni è stato accostato a questo disegno di legge. Presidente, questo è e sarà il modello italiano del Governo Meloni, del ministro Bernini e del Parlamento italiano. Inoltre è importante precisare che i ragazzi potranno seguire il loro primo semestre in qualsiasi ateneo, perché i programmi saranno i medesimi, e che quelli selezionati in base alla loro posizione nella graduatoria unica nazionale decideranno dove continuare a studiare, esattamente come avviene oggi, esprimendo preferenze. Anche qui ci sarà quindi un risparmio per le famiglie e non un aggravio, come qualcuno dell'opposizione ha ipotizzato. Presidente, piuttosto tanti interventi, spesso senza nessuna attinenza all'oggetto del disegno di legge (scuole di specializzazione, trattamento economico dei medici, organizzazione del servizio sanitario, qualità dell'assistenza medica), con proclami catastrofici, in modo particolare da parte dei colleghi del PD, mi portano a pensare che o non hanno letto il testo o hanno letto - forse in modo più conveniente per loro - qualche lettera che proveniva da qualche sindacato, peraltro male informato.

per questo desidero ringraziare ancora una volta il ministro Bernini, per la grande attenzione che sta dimostrando su questo tema, visto che è stato già costituito un tavolo di lavoro sulla riforma che suggerirà la scelta delle discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre e il metodo da adottare per valutare il superamento dei relativi esami. Su questi punti Fratelli d'Italia ritiene che l'anatomia, per esempio, debba essere una materia caratterizzante fondamentale, anche per facilitare il percorso di auto-orientamento dei ragazzi, e che il sistema migliore per la selezione al termine del semestre sia una valutazione nazionale uguale per tutti, che assegni un voto per ogni disciplina e quindi determini una graduatoria equa, garantendo assoluta parità di condizioni. Ribadisco che abbiamo assoluta fiducia nel Ministro e nel suo operato. Concludo, Presidente. Fratelli d'Italia è convinta che con l'attuale riforma proposta si investa realmente sul futuro dei nostri giovani, garantendo in modo efficace l'opportunità di perseguire, ad armi pari per tutti, il sogno di diventare medici. Non solo: si investe sul futuro della nostra Nazione, favorendo l'accesso alla facoltà di medicina dei più meritevoli, pur mantenendo nel lungo corso di laurea una formazione di qualità e un'offerta formativa d'eccellenza. Per questi motivi sono fiera di dichiarare il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

oggi voglio portare a conoscenza dell'Assemblea un gravissimo fatto che sta accadendo in provincia di Cuneo, più precisamente a Santa Vittoria d'Alba, dove la multinazionale britannica Diageo, colosso mondiale nel settore delle bevande alcoliche, ieri ha annunciato la chiusura entro giugno 2026, dello storico stabilimento ex Cinzano. Una decisione comunicata purtroppo a bruciapelo, con una lettera ai 349 lavoratori, lavoratori, gettando in ginocchio loro, le loro famiglie e colpendo al cuore tutta la Provincia Granda. La lettera è arrivata pochi giorni dopo l'informativa in cui le parti sindacali, mostravano preoccupazione sulla situazione in cui versa il sito produttivo di Santa vittoria d'Alba. La ex Cinzano, dal nome della frazione in cui sorge la fabbrica, è un'azienda storica, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, uno dei tanti preziosissimi simboli dell'Italia che lavora e crea prodotti di grandissima qualità. La prospettata chiusura è una ferita per tutto il *made in Italy*. In quello stabilimento si è scritto un pezzo importante della storia dell'"Italia da bere"; da lì il marchio Cinzano conquistò il mondo della moda e dello sport. La Diageo gruppo è quotata La Diageo gruppo è quotata alla borsa di Londra, è presente in 180 Paesi al mondo, con oltre 200 prodotti. L'unico sito produttivo in Sud Europa si trova proprio in Italia, a Santa vittoria d'Alba. L'azienda nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2024 ha comunicato un fatturato di vendite nette pari a 20,3 miliardi e un utile operativo che ha raggiunto i 6 miliardi di euro. Insomma, noi non stiamo parlando di una multinazionale in crisi, anzi; questa realtà e il suo valore produttivo vanno tutelati e con essi le centinaia di posti di lavoro che continua a offrire sul territorio. La procedura di consultazione con i sindacati è già stata avviata ed oggi le segreterie provinciali di Fai CISL, Flai CGIL, UILA, UIL e UGL, hanno indetto uno sciopero di otto ore per ogni turno di lavoro. L'azienda, dal canto suo, ha fatto sapere di essere disponibile per esplorare soluzioni alternative per il futuro. Anche le istituzioni hanno il dovere di intervenire per fermare tutto questo e dare risposte al territorio. Oggi dunque chiedo, tramite lei, Presidente, l'attenzione del Governo su questa delicatissima vicenda in quanto non si può permettere a un'azienda di questo calibro di chiudere uno stabilimento in Italia, lasciando per strada 349 persone con le loro famiglie. Chiedo anche quali interventi sarebbe possibile attuare a livello di Ministero delle imprese e del *made in Italy* e di Ministero del lavoro per difendere la fabbrica, i lavoratori e con essi una parte importante del *made in Italy*. Oggi ho presentato un'interrogazione qui in Senato, nella quale oltre ad una particolare attenzione a questo drammatico evento, chiedo anche l'istituzione immediata di un tavolo di concertazione presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con tutti i soggetti coinvolti al fine di analizzare da subito la problematica e trovare la soluzione più favorevole per la continuità dell'attività dell'impianto produttivo e il mantenimento dell'occupazione. *(Applausi)*.

che è una risposta che proprio non si regge in piedi, incongruente e contraddittoria. Va bene che il Parlamento interroghi il Governo, ma il Governo poi deve dare delle risposte che reggano. Cerco di spiegare la situazione. L'interrogazione si riferiva a un nostro ex collega, Stefano Esposito, che è stato intercettato mentre era membro del Parlamento, precisamente era senatore, più di 500 volte ed è stato poi rinviato a giudizio, sulla base di 130 di queste intercettazioni che erano state recepite tutte senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza. Viene sollevato conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale e quest'ultima, nel dicembre del 2023, censura pesantemente la procura di Torino per aver utilizzato illegittimamente delle intercettazioni del senatore Esposito. Ora, queste intercettazioni, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, dovevano essere distrutte perché erano state - ripeto - illegittimamente percepite. Accade, però, che improvvisamente queste intercettazioni vengono fuori in un fascicolo di causa che non riguarda neanche il collega Esposito, dove lui non è neanche imputato, quindi delle intercettazioni che dovevano essere distrutte riaffiorano in un fascicolo di causa e vengono di nuovo rese pubbliche senza che Esposito A questo punto, chiedo al ministro Nordio di farmi capire cosa sta succedendo e se intende mandare degli ispettori alla procura di Torino. Nordio mi risponde non di aver mandato gli ispettori, ma di aver chiesto alla procura di Torino di dirgli che cosa era successo e quindi mi dice che cosa è successo, ma le spiegazioni proprio non si reggono. Cosa dice

imputati, le intercettazioni sarebbero spuntate nel fascicolo. Questa spiegazione non regge, in primo luogo perché gli atti tornati indietro non riguardano Stefano Esposito, perché Stefano Esposito non è imputato in quel procedimento, quindi la cosa non ha senso; in secondo luogo, perché Torino, a suo tempo, mandò a Roma le trascrizioni, ma non le fonie, cioè non i nastri registrati: quei nastri registrati non si sono mai mossi da Torino. Quello che vorrei capire, allora, è se li hanno distrutti o

che non siano rilevanti è fuori discussione, perché Esposito - ripeto - non è imputato in quel procedimento. Invece posso affermare - ed è qui che quindi trovo un elemento di falsità materiale nella risposta che il ministro Nordio mi dà e il Ministro non può mentire al Parlamento, perché mi dice che queste intercettazioni non ci sono - che ci sono 60 di queste intercettazioni nel faldone numero 13 del procedimento. Le cose non funzionano perché se un parlamentare fa una domanda, il Ministro deve rispondere la verità; se il Ministro si è fidato della procura di Torino e mi ha fatto rispondere cose che non stanno né in cielo né in terra, allora sarà bene che il Ministro mandi finalmente degli ispettori alla procura di Torino, perché se quando loro rispondono poi mi dicono queste cose che non stanno in piedi, forse varrebbe la pena che il Ministero della giustizia mandasse qualcuno dei suoi a Torino a vedere che cosa succede, perché una procura che intercetta per 500 volte un parlamentare senza chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza e poi non distrugge gli atti che la Corte costituzionale le ha detto di distruggere, quanto meno suscita qualche perplessità e qualche interrogativo a cui bisognerebbe dare risposta attraverso l'ispezione. Per suo tramite, signor Presidente, chiedo pertanto agli uffici di inviare la trascrizione di questo mio intervento di fine seduta al Ministero della giustizia perché proceda di conseguenza.